Presidente, desidero segnalare alla Presidenza un fatto che a mio avviso assume una sua particolare gravità. Oggi, nel corso della seduta della Commissione affari costituzionali, abbiamo appreso

che questo tempo è assolutamente ridotto rispetto alla serietà e alla gravità dei problemi. Noi dell'opposizione intendiamo legittimamente portare, in maniera pacata, garbata e serena la nostra voce, nel tentativo di migliorare questo decreto. Lei capisce, però, che in tre ore questo non è possibile, specialmente alla luce della circostanza, signor Presidente, che leggiamo sul giornale

ma noi siamo costretti a discutere su un decreto-legge che, sulla base di dichiarazioni ufficiali di autorevoli esponenti del Governo e della maggioranza, ci appare essere superato. In sintesi, signor Presidente, la pregheremmo di voler intervenire per consentire un allargamento dei tempi del dibattito e conseguentemente consentire ai senatori dell'opposizione di poter partecipare in maniera seria e costruttiva alla costruzione di un decreto che non deve corrispondere alle esigenze di una parte politica, ma solo ed esclusivamente, nell'ambito della legalità, alle esigenze di sicurezza dei cittadini.

Siccome il decreto‑legge sulla sicurezza contiene numerose, significative e determinanti disposizioni di tipo giurisdizionale e siccome la Commissione giustizia, della quale faccio parte, intende occuparsene molto seriamente e molti dei colleghi intervenuti di fatto chiedono che il decreto

sulle espulsioni non è stato ancora presentato né alla Camera né al Senato, non sapremmo di cosa dobbiamo discutere. O il decreto‑legge è la riproposizione del disegno di legge e ha un significato, o è un'altra cosa e ha un altro significato. È una questione che attiene ragionevolmente ai tempi dell'esame, che in in Commissione giustizia vorremmo che fossero un po' più ampi, non per fare ostruzionismo, ma perché dobbiamo capire se il decreto può essere lasciato cadere perché vi è un disegno di legge oppure Se il disegno di legge non è ancora stato presentato a nessuna delle due Camere, vorrei capire dal Governo e dal Ministro della giustizia di che cosa stiamo discutendo. Dal momento che era presente il sottosegretario Scotti e non il ministro Mastella, ricordo che si del rapporto tra Parlamento e Governo. Non è solo questione di tempo, come ha detto il collega Nitto Palma, ma è una questione decisiva di ordine costituzionale. Desidero che il ministro Mastella ci faccia sapere

per scusarmi con lei in quanto ieri, in maniera, spero, mai poco garbata, le ho richiesto più volte per quale motivo non avessi la parola. Un funzionario mi ha spiegato che precedentemente era stato

Presidente, vorrei rispondere alla questione posta con il consueto garbo e con la pacatezza che gli riconosciamo dal collega Palma, anche se obiettivamente debbo dire che poteva e può essere posta nella sede propria, che è quella dell'Ufficio di Presidenza della Commissione affari costituzionali, della quale il collega Palma è vice presidente. Se il collega Palma fosse stato presente alla riunione avrebbe saputo perfettamente che non ci è stata imposta alcuna limitazione a tre ore del dibattito in Commissione affari costituzionali. Addirittura io, come Presidente, avevo chiesto di prevedere una sessione per lunedì ed è stato il collega Calderoli a suggerire che, poiché si poteva discutere martedì, mercoledì e anche giovedì, appariva

non vedo la questione nei termini espressi, con qualche sottolineatura polemica, da parte del presidente D'Onofrio.

da ciò a ritenere che un decreto-legge presentato debba essere fatto cadere dal Governo, francamente non mi sembra questo l'esercizio che in questo caso il Governo vorrebbe porre in essere nei confronti della Commissione cui ella ha fatto riferimento.

Signor Presidente, intervengo per annunciare il voto contrario su questo emendamento, pur riconoscendo che le questioni a cui esso

quindi, produce un contributo importante al fabbisogno energetico della Nazione. D'altro canto, però, a noi non deve sfuggire che, quando si tratta di questioni riguardanti l'uso delle risorse e le politiche energetiche, bisogna sempre aver presente quali siano gli interessi nazionali, le compatibilità generali e gli effetti che le soluzioni, che di volta in volta si presentano, possono portare a questa scelta e a questo indirizzo. Non c'è dubbio che esista, comunque, un problema relativo ad una migliore sistemazione del rapporto tra la Regione, che è la maggiore tributaria

già da tempo ci si muove in questo senso. Vorrei che noi potessimo affrontare questo tema in un quadro di minore - se mi è concesso dirlo - episodicità ed estemporaneità, qual è un emendamento alla legge finanziaria, di un ripensamento organico dei rapporti tra la Basilicata e il resto del Paese per quanto riguarda la disciplina degli interventi relativi all'utilizzazione delle sue risorse energetiche. Infatti, non sono del tutto certo, per esempio, che una compensazione passante attraverso la riduzione delle accise alle pompe di benzina o di gasolio

Mi verrebbe da dire che, se noi perseguissimo questa strada, per quanto mi riguarda avrei molti meno argomenti per controbattere al ragionamento fatto, ad esempio, stamattina dal senatore Castelli in merito al fatto che le erogazioni fiscali che l'Italia del Nord offre al Paese dovrebbero, in termini di servizi, ritornare per

una politica delle perforazioni che intervenga in maniera indiscriminata su tutto il territorio regionale. Da questo punto di vista non ho sicurezze: non so quando sia opportuno fermarsi, in Basilicata, nel dare concessioni di estrazione alle società petrolifere; è però certo che ormai in quella Regione si sta sviluppando un movimento di opinione pubblica che ritiene che si sia giunti al punto limite e che non si possa fare della Basilicata, sostanzialmente, una Regione tutta segnata da attività dell'industria estrattiva.

ma anche per sostenere convintamente le ragioni che pretendono di effettuare una profonda modifica di tutto il sistema delle accise e della loro attribuzione ai diversi livelli di responsabilità di governo nel nostro territorio. La Regione Basilicata, Regione produttrice, ha il giusto diritto di vedersi riconosciuta una quota importante di quell'introito, che è parte delle casse dello Stato, sia direttamente

nella scorsa finanziaria, era già intervenuto disciplinando la materia, seppure in modo parziale, e relativamente a un comma della legge finanziaria che riguardava

- la "retrocessione" (ma io voglio definirlo come "riconoscimento") di una quota delle accise alla Regione come elemento compensativo per l'incremento della quota di compartecipazione alla spesa sanitaria. Quella vicenda costituisce una lesione delle prerogative parlamentari, perché quella norma, perfettamente approvata secondo la ritualità del Parlamento, è stata pervicacemente ignorata, disapplicata, contestata dai comportamenti del Ministero dell'economia che, per così dire, non soltanto ha preteso di reinterpretarla in linea amministrativa, ma in una serie di occasioni, sia a livello di burocrazia che a livello di responsabilità politica, si è anche permesso di contestare l'autorità del Parlamento a interferire in materia. Avevo presentato un emendamento che riproponeva la questione in termini, per così dire, ancor più marcati e complessivi, prevedendo l'intera attribuzione della responsabilità alla Regione della spesa sanitaria e di altre funzioni che potevano ad essa essere trasferite sulla base del principio di simmetria, ovviamente avendo un riconoscimento sul gettito (quota o complessivo) delle accise del prodotto pertrolifero raffinato nelle Regioni Sicilia, Sardegna ed altre, dove insistono impianti di raffinazione. Inoltre, signor Presidente, accanto alla questione Basilicata dell'attività estrattiva, vi è un'altra gravissima questione che riguarda gli impianti di raffinazione, per la grandissima parte insediati in Sicilia e Sardegna, che determinano gravissimi danni ambientali oltre che comprovati danni alla salute emersi da rigorosissime ai quali non deriva alcun beneficio al territorio in cui quegli impianti insistono. In una logica di federalismo fiscale

di questi introiti sulla base di attribuzione di competenze: non vogliamo benefici a poggia, vogliamo una revisione del sistema delle accise in cambio dell'assunzione delle responsabilità di competenze. L'anno scorso questo era avvenuto, il Parlamento ha votato un emendamento della maggioranza, il Governo ha disatteso, ciò costituisce una lesione statutaria e anche delle prerogative parlamentari. Il mio emendamento è stato giudicato inammissibile dalla Commissione bilancio, ne ho chiesto formalmente la riproposizione, non lo trovo inserito

e non vorrei che fosse frainteso come un atteggiamento di lesina da parte dello Stato nei confronti di una Regione tradizionalmente una piccola Regione come la Basilicata, che è stata già depauperata da una industrializzazione abortita e fallita negli anni Sessanta (ricordo lo sfacelo dell'ENI e della chimica pesante) e ha subito una trasformazione del territorio terribile,

e purtroppo dobbiamo constatare come la questione petrolio renda spesso la classe politica lucana subordinata nella gestione della cosa pubblica rispetto a questa ricchezza. Soltanto i partiti del centro-destra sono estranei a questa logica del potere, che ha visto incollate nei microcosmi dei paesi lucani classi che si sono succedute attraverso una gestione ormai cinquantennale del potere, e a questo sfruttamento delle risorse petrolifere che, incidendo sul territorio dal punto di vista morfologico, hanno fatto sì che la Regione Basilicata non sia più il polmone verde del Sud d'Italia, ma nello stesso tempo ha permesso a chi detiene il potere di sfruttarla in maniera servile, senza guardare agli interessi generali. Ecco perché l'emendamento 3.0.2 costituisce un modesto segno di attenzione, che va coltivato, va ampliato, va amplificato, se vogliamo far sì che nel Sud d'Italia si redistribuiscano le ricchezze in maniera paritaria e uguale.

ma non entra né nel merito delle questioni sollevate circa l'eccessivo sfruttamento della Regione Basilicata in termini di estrazione di prodotti gassosi e petroliferi, né nel criterio di proposizione e formulazione dell'emendamento. Ciò che alla Lega interessa di questo emendamento

Non potrà essere uno sconto sulla benzina a risarcire i cittadini lucani dai danni che già oggi le estrazioni petrolifere producono in termini di ricadute sulla qualità dei prodotti agricoli, dell'aria e sulla possibilità di una elevata

che puntino sulla valorizzazione delle risorse della nostra terra, a partire da un'agricoltura e da un turismo di qualità, da innovazioni tecnologiche in campo ambientale, da politiche di risparmio energetico e di energia alternativa. modelli, lavorando in sinergia con le università e gli enti di ricerca, potrebbero dare una prospettiva nuova ai giovani laureati lucani che oggi, come negli anni Sessanta, abbandonano ed emigrano dalla nostra terra.

**Il Senato non approva.**

un contenuto piuttosto esigente giacché immagina di attivare un meccanismo di fiscalità differenziata per le imprese attraverso una norma della finanziaria, per me l'occasione per riportare all'attenzione di quest'Aula una questione che è sempre condivisa nell'ambito delle riflessioni teoriche, nei seminari e nei confronti rilassati del ragionamento politico, ma che non trova mai la possibilità di tradursi in un'iniziativa concreta. Qualche mese fa, durante il dibattito sul Documento di programmazione economico-finanziaria, avevo introdotto una previsione una previsione affinché in quel documento (che quindi definisce le linee della programmazione e non è un atto vincolante dal punto di vista normativo) vi fosse un orientamento del Governo volto a sperimentare meccanismi di fiscalità compensativa nelle aree ad Obiettivo convergenza.

sulla base di un'intuizione condivisa secondo cui i meccanismi di sviluppo che devono assistere la crescita del Mezzogiorno devono essere ricercati negli automatismi e non negli incentivi, ho riproposto la necessità di una scelta di sistema attorno alla fiscalità di vantaggio. Cosa trovo in questa finanziaria? Trovo un intervento importante sulla fiscalità per le imprese, sull'IRES e sull'IRAP, ma in modo totalmente indistinto sul territorio nazionale. Ciò vanifica la possibilità di attribuire un vantaggio competitivo alle aree di maggior disagio sia per ragioni infrastrutturali, sia per ragioni di marginalità geografica, nonché per condizioni sociali ed economiche. Questo Governo e questa maggioranza, al di là del fatto che declinano tale possibilità in termini puramente teorici, in condizione di affrontare il tema dello sviluppo in linea con le indicazioni e gli orientamenti di Bruxelles? Nell'emendamento 3.0.3, a mia firma, si fa riferimento ad un'indicazione quale si comincia ad ammettere la possibilità di una fiscalità differenziata nelle aree dell'Obiettivo convergenza, ma debbo registrare che perfino l'intuizione riduttiva, per non dire micragnosa, delle zone franche urbane non è stata attivata. È stata introdotta una norma inapplicabile e, tra l'altro, assistita da una dotazione finanziaria assolutamente inconsistente. Allora vi chiedo,

attribuzioni e risorse conferite attraverso la mediazione politica, ma meccanismi automatici che bonificano anche il rapporto tra politica e territorio. È una scelta innovativa ed è l'unica che ha un senso

quel processo di avviamento e quel percorso di valorizzazione delle Regioni che si può attuare anche con la riscossione diretta dell'IRAP.

dei propri esattori, un controllo diretto sul territorio e un rapporto più civile con il contribuente è un passo necessario in direzione del federalismo fiscale.

che percepiscano un reddito, proprio e del coniuge, non superiore a 516,46 euro per 13 mensilità (e cioè il vecchio milione di lire), a condizione che non vi siano altre persone conviventi e che l'apparecchio sia ubicato nel loro luogo di residenza. Si tratta di cittadini che versano in condizioni economiche estremamente precarie, che hanno nello strumento televisivo l'unica possibilità di tenersi informati e di trovare un minimo di svago: per essi il pagamento del canone rappresenta una spesa assolutamente insostenibile. vogliamo ringraziare i colleghi Zanda, Peterlini e Formisano, che hanno ritenuto di aggiungere la loro firma al nostro emendamento; ringraziamo fin d'ora anche gli altri colleghi che vorranno fare altrettanto. nel fatto che l'Aula possa approvare all'unanimità questo nostro piccolo, ma grande emendamento.

il parere è favorevole, pur nella consapevolezza - lo dico all'Aula, prima che si diffonda un'opinione diversa - che si tratta di un gesto, appunto, molto significativo,

di una coppia di anziani con un reddito inferiore a 516 euro al mese. Sarà, quindi, una platea molto contenuta, però, è un gesto significativo. qui c'è un problema di quantificazione, su cui mi rimetto al Governo, e c'è un problema di applicazione concreta della norma, per la quale si prevede il rinvio ad un decreto ministeriale che dovrà essere emanato. GRANDI,

è molto difficile fare una quantificazione in tempo utile, ed è la ragione per cui si è preferito in questo momento mettere la posta in bilancio; vedremo poi se vi saranno le condizioni per avere un allargamento del finanziamento, giacché ovviamente non potremo lasciare una parte di anziani con e una parte di anziani senza, ma in questo momento non siamo in grado di fare una previsione più corretta. In secondo luogo, sono d'accordo con anche se la valutazione non è ancora pronta e quindi in questo momento lo faccio senza prendere impegni né in un senso né nell'altro.

che danno in molti casi agevolazioni molto forti alle imprese (in questo caso, ripeto, a piccolissime imprese), mentre per i lavoratori, e per quelli dipendenti in particolare, ci sono solo gli ordini del giorno o le promesse di un contributo futuro. Registro che ancora una volta si procede in questo modo.

Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del Gruppo Sinistra Democratica. Qualche giorno fa, come i colleghi ricorderanno, un orientamento favorevole in tal senso era stato espresso dal senatore Brutti alla fine di una riunione della Commissione bilancio. Anche i giornali autorevolmente ne avevano dato notizia. Quindi, non possiamo che essere d'accordo con un emendamento di questo tipo. auspichiamo che possa estendersi ulteriormente la platea degli anziani soli con pensione minima e che il provvedimento nel futuro possa riguardare altri servizi che non siano solo quelli radiotelevisivi.

*bipartisan* al fine di alleviare i problemi che in questo momento soffrono i pescatori, dovuti all'aumento del costo del petrolio e quindi del gasolio. Lei sa, signor Presidente, che era stata prevista una disposizione a favore dei pescatori con uno stanziamento di 12 milioni di euro per allargare la platea dei beneficiari della cosiddetta IVA speciale agricola anche ai pescatori. Nonostante gli sforzi, bisogna darne atto, del ministro De Castro presso la Commissione europea, questa non ha tuttora autorizzato lo Stato italiano

il caso di non perdere questi 12 milioni di euro. Ho quindi proposto, signor Presidente, di elevare dal 70 all'80 per cento i benefìci previsti dalla legge n. del 1998, cioè gli sgravi fiscali contributivi a favore della pesca costiera e lagunare. In questo modo eviteremo che 12 milioni di euro a favore dei pescatori italiani,

senza nuovi costi, senza maggiori oneri, evitando che 12 milioni di euro vadano in perenzione.

Troppo spesso è accaduto nel nostro Paese, e anche in questa legislatura, che una retroattività insieme ad un'incapacità o ad un'impossibilità da parte delle aziende di valutare l'azione di revisione degli studi di settore nell'esercizio già iniziato, inoltrato o addirittura già finito,

ma rende stabile l'applicazione dello statuto del contribuente, nel momento in cui non prevede una retroattività, che a questo punto non deve valere solamente da un esercizio ad un altro, ma anche all'interno dello stesso esercizio: le rivalutazioni degli studi di settore debbono iniziare ad avere effetti concreti dall'esercizio successivo entro il quale sono state attuate.

una previsione fatta nella scorsa finanziaria per alcune zone del Paese. Sto parlando dell'attribuzione di zona franca, che era stata stabilita con delle peculiarità specifiche nella scorsa legislatura e che questo emendamento estende a tutti i Comuni confinanti con Paesi esteri o con le Province o Regioni autonome, che hanno una fiscalità

cui confini si trovano delle situazioni diverse e privilegiate in ordine alla fiscalità: sappiamo quanto sia diversificato questo aspetto soprattutto fra il Veneto e l'Alto Adige o fra la Lombardia il Trentino oppure fra il Veneto ed il Friuli. Sappiamo che, passando questi confini - che stanno diventando mitici - gli imprenditori e i cittadini possono usufruire di servizi in qualità ed in quantità enormemente superiori. È evidente che questo *gap* non può essere superato in pochi giorni o in pochi mesi, finché in questo Paese non ci si deciderà finalmente a dare concretezza ad un federalismo vero e che comprenda nei suoi aspetti tanto quello politico-amministrativo, quanto quello fiscale. sarebbe un sistema per dare una risposta. Qual è la risposta che daranno queste Aule parlamentari quando arriveranno i disegni di legge relativi al trasferimento, ad esempio, dell'Altopiano di Asiago al Trentino o della zona

posizione seria e valida, avremo dato una risposta a dei problemi o avremo solo fatto finta - che si dia una risposta affermativa o negativa - che questi problemi non esistano? È solo con un'azione

questi sono plebisciti veri, di persone, di cittadini stanchi di avere una situazione fiscale totalmente diversa e svantaggiata, che vogliono staccarsi dalle Regioni; il risultato della mancata risposta di questo Stato all'esigenza di autonomia e di federalismo, di essere, per lo meno nei confronti dei dirimpettai, simili e paragonabili quanto a disponibilità di risorse e di risposte che chiedono ovviamente i propri cittadini. Questo dice l'emendamento 5.91, che tratta tratta la questione in un suo aspetto peculiare, marginale e specifico, quello di creare delle zone franche in questi Comuni e che non ha la pretesa di dare la risposta vera ed autentica di federalismo, ma è comunque un emendamento che prende in considerazione le esigenze espresse dai cittadini.

da questo emendamento. Invito, quindi, tutti i colleghi, prendendo spunto dall'iniziativa che era stata assunta da questa maggioranza nella finanziaria scorsa, a prendere in considerazione un voto positivo su questo emendamento. *(Applausi

5.106 sull'abolizione della possibilità di installare gli apparecchi da gioco nelle sale Bingo. Signor Presidente, Cavour diceva che il gioco è la tassa sui poveri.

Il presidente dell'Antimafia Forgione ha affermato: «È evidente che la circolazione di contanti senza controllo alcuno e la facilità di riciclare all'interno di queste gestioni rischiano di creare un corto circuito pericoloso che va interrotto». Un'ambiguità che viene segnalata e rimarcata anche dalle indagini delle procure di Biella

è una percentuale statistica enorme di persone affette da disturbo da dipendenza nel nostro Paese. Nella Provincia di Varese si calcolano tra le 5.000 e le 7.000 persone affette da gioco dipendenza patologica. È evidente che vi sono le prove provate le prove provate di connessioni tra il gioco delle macchinette, la mafia e anche connivenze politiche che poi, magari, verificheremo. oggi la possibilità di installare le macchinette anche nelle sale Bingo significa fare un regalo, abbastanza evidente, alla zona di ambiguità che contraddistingue questo settore.

che consenta alle aree di confine della Regione Friuli-Venezia Giulia di competere con la Slovenia. Ho chiesto al Governo e al relatore la possibilità di effettuare un approfondimento tecnico e quindi di accantonare l'emendamento

Abbiamo presentato cinque emendamenti all'articolo 5 che fanno riferimento alle problematiche che ineriscono agli studi di settore.

come questa non si può improvvisare per raggiungere gli obiettivi che noi auspichiamo. Abbiamo voluto segnalare che sugli studi di settore si apre, per quanto riguarda i senatori della Costituente Socialista, la

ora. A nostro giudizio, infatti, è venuto il momento perché si stabilisca, in coerenza con tanti atti che il Parlamento ha prodotto, con mozioni che

strumenti di coercizione o di imposizione, ma di orientamento nell'accertamento del reddito delle categorie interessate. Per questo noi teniamo particolarmente all'avvio di questa riflessione; tuttavia, comprendendo

*Dopo il comma 74, è inserito il seguente:* «74-*bis*. All'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il primo periodo, inserire i seguenti: "Ai fini dell'accertamento l'Agenzia delle entrate ha l'onere di motivare e fornire elementi di prova per avvalorare l'attribuzione dei maggiori ricavi o compensi derivanti dall'applicazione degli indicatori di normalità economica di cui al presente comma, approvati con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 20 marzo 2007, sino alla entrata in vigore dei nuovi studi di settore varati secondo le procedure, anche di concertazione con le categorie, della In ogni caso i contribuenti che dichiarano ricavi o compensi inferiori a quelli previsti dagli indicatori di cui al presente comma non sono soggetti ad accertamenti automatici."». Questa è, dunque, la nuova formulazione che abbiamo concordato, che sottoponiamo alla valutazione del relatore e del Governo e su cui ci esprimeremo in sede di dichiarazione di voto - lo farà il presidente Angius - per valutare l'atteggiamento del Governo e del relatore. Colgo l'occasione, signor per dire che mi sembra sensata la proposta, avanzata prima di me dal senatore Antonione,

Stiamo parlando di una proposta di modifica che riguarda la disciplina prevista dai commi dal 41 al 46 sulle disposizioni in materia di fatturazione elettronica.

7 marzo 2005, n. 82, in ottemperanza ad una direttiva europea del 2001. È stato un percorso lungo, perché occorre arrivare alla rivoluzione digitale e consentire che finalmente ogni tipo di fatturazione nel rapporto con il servizio pubblico sia legata all'elettronica ed alle opportunità offerte dall'informatica. L'avvertimento di carattere tecnico, relatore, è che il comma 42 fa riferimento ad un regolamento previsto dal

rapido che si vuole qui introdurre, che rischia di andare a scapito di un corretto funzionamento del sistema. Mi spiego meglio: con questa norma prevediamo che, a partire dall'entrata in vigore di quello che si chiama regolamento da una parte e decreto dall'altra,

ad un sistema che si intende rivoluzionare e che per la fretta (rendiamoci conto che qui partiamo dal 2001; il percorso non è stato lento, ma ha avuto i sui tempi: 2001, 2004, 2005) rischia di fare,

che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento, non si possa procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, fino all'invio in forma elettronica. Questo rischia di danneggiare colui il quale invece si vorrebbe favorire con un meccanismo trasparente. Raccomando dunque al relatore attenzione sull'emendamento che mi sono permesso di proporre, che serve a migliorare una norma giusta. Mi raccomando anche di verificare in sede di coordinamento

richiamando in particolare l'attenzione del relatore, senatore Legnini, del presidente della Commissione, senatore Morando, ed anche di tutti i colleghi eletti in Liguria, Lombardia, Piemonte e Friuli-Venezia Giulia. Nella finanziaria è stato Nella finanziaria è stato introdotto un principio che ci trova consenzienti; un principio, se volete, assai positivo che potremmo enfaticamente definire l'inizio di un federalismo portuale. portuale. Nella norma proposta dal Governo si dice che l'extragettito, cioè ciò che in più arriverà nella movimentazione dei traffici portuali in termini di tasse che si pagheranno sull'imbarco e lo sbarco delle merci, potrà essere utilizzato dalle Regioni di riferimento del territorio per fare opere pubbliche stradali, autostradali e ferroviarie.

si è avuta notizia che il Governo ha fatto questa proposta, nelle singole Regioni, a livello di Province, di Comuni e di enti locali

che, sforzandomi, ho scoperto in questa proposta di finanziaria. Vorremmo soltanto che le risorse da quantificare venissero più precisamente finalizzate per realizzare le opere pubbliche. A casa mia, a Genova, in Liguria, ovviamente il riferimento è al terzo valico, cioè all'opera strategica più importante per il futuro della Regione Liguria e di quell'area vasta considerata il Nord-Ovest del Paese, cioè il retroterra del porto di Genova,

con i porti adeguatamente organizzati potrà far crescere una movimentazione del traffico delle navi provenienti dall'estremo Est, con quello che sta avvenendo sul mercato cinese ed indiano. Per questi motivi, signor Presidente, richiamo l'attenzione dei colleghi eletti in questa Regione, perché mi pare una norma di miglioramento rispetto ad un principio su cui siamo d'accordo.

che quindi occorressero risorse aggiuntive. Pur tuttavia, per accogliere la sollecitazione del senatore Scarpa Bonazza Buora, dopo aver ascoltato gli argomenti che egli ha

caso preannuncio che sarei favorevole, tanto più che questo testo era già stato presentato anche dagli altri colleghi della Commissione di merito e poi è stato ritirato per questa stessa ragione. Quindi, sono d'accordo

5.31 vi è una richiesta di accantonamento; riguarda il cosiddetto pacchetto Friuli. Il Governo aveva fatto una valutazione, pervenendo ad un

copertura che non comporti attingimento di risorse rilevanti. Inviterei il Governo, nell'aderire all'accantonamento, ad una più puntuale valutazione del testo.

Nella mia breve esperienza di pochi mesi nella passata legislatura ricordo le battaglie che su questo problema fece il senatore Pizzinato;

ove l'emendamento fosse accolto, di determinare una finalizzazione ben precisa delle risorse aggiuntive per le infrastrutture. Questa finalizzazione può essere condivisibile, ma forse sarebbe più opportuno lasciare alle Regioni l'autonomia decisionale di stabilire a quali infrastrutture destinare quelle risorse aggiuntive. Per tale ragione il parere è contrario.

finalizzato ad introdurre un principio di grandissimo rilievo, vale a dire che gli indicatori di normalità economica, che sono stati definiti sulla base della normativa dello scorso anno, costituiscono presunzioni semplici ovvero che l'onere della prova relativamente al mancato rispetto degli indicatori di normalità spetta all'amministrazione finanziaria. quella norma viene ulteriormente rafforzata ed esplicitata, soprattutto in relazione alla sua vigenza sotto il profilo temporale: vale, quindi, fino a quando non verranno ridefiniti gli studi di settore con le categorie interessate.

dell'emendamento 5.69 destrutturerebbe l'intero sistema degli studi di settore, con una potenziale perdita di gettito di enorme rilevanza. È evidente, pertanto, che una proposta di tal genere non è accoglibile. Per inciso, faccio notare al senatore Azzollini e ad altri senatori che neanche il loro Governo si è azzardato ad osare tanto, cioè a considerare tutti gli studi di settore come presunzioni semplici.

di spostare 12 milioni di euro (appostati già nella Tabella 13 del Ministero dell'agricoltura, per far fronte all'IVA agricola, che non può essere applicata alla pesca, in quanto non siamo autorizzati da Bruxelles), aumentando

È meglio dire subito se si è favorevoli a non perdere soldi a favore dei poveri pescatori o se si preferisce perderli e farli andare in perenzione.

la norma che proponiamo ‑ lo ribadisco ‑ non costa alcunché. Abbiamo apprezzato l'iniziativa del Governo che con questa finanziaria avviato un principio molto importante, che potremmo definire di federalismo portuale. Siamo, quindi, d'accordo sulla norma contenuta al comma 70 dell'articolo 5. Semplicemente, abbiamo registrato osservazioni quantomeno originali e strane nella recente assemblea di ASSOPORTI, dove pare che i più e i tanti si siano adoperati per correre sopra al carro e in qualche modo proporre utilizzi strani e originali di questo extragettito. pertanto che il Parlamento si pronunciasse finalizzando in modo puntuale le risorse che proverranno alle Regioni in virtù di un maggiore incremento della movimentazione portuale, a favore delle opere pubbliche strategiche. Queste ultime sono quelle di cui alla delibera del 21 dicembre 2001, i cosiddetti corridoi plurimodali, che interessano il porto di Genova, quindi tutto l'*hinterland* del Nordovest, il porto di Trieste, quindi la Padania, Grazie, come hanno suggerito il relatore ed il Governo, allora si deve sapere che da domani siamo autorizzati a recarci sui territori di riferimento a dire che questa maggioranza è condizionata da forze di un certo tipo, che non credono alle opere strategiche di cui alla delibera del 21 dicembre

pur avendo risorse potenzialmente disponibili e il consenso del territorio (perché il Corridoio del terzo valico ha avuto l'approvazione delle Regioni Lombardia, Liguria e Piemonte e di tutti i Comuni interessati), in realtà, alla prova provata, non si accetta questa proposta di finalizzazione e si vota contro.

**Il Senato non approva.**

**Il Senato non approva.**

della ordinaria procedura di consultazione delle organizzazioni rappresentative del lavoro autonomo, introducendo quegli indicatori di normalità ai quali era stato dato un effetto retroattivo, nel senso che essi avevano modificato gli studi di settore con la conseguenza dell'inversione dell'onere della prova nel caso di scostamento dei contribuenti dagli studi stessi. In quell'occasione, furono votate più mozioni, in particolare il Senato approvò una mozione

uno strumento di ausilio e supporto per compiere le attività di controllo ed accertamento della regolarità delle dichiarazioni da parte dell'amministrazione finanziaria, in una logica che in modo inequivocabile respinge ogni forma di catastizzazione o di reintroduzione surrettizia della *minimum tax*»". In sostanza, la mozione di maggioranza diceva inequivocabilmente che gli studi di settore non devono rappresentare una soglia obbligatoria minima di reddito al di sotto della quale collocandosi il contribuente scatterebbe l'inversione automatica dell'onere della prova.

di normalità deve avvenire con l'ausilio irrinunciabile delle associazioni di categoria interessate, restituendoli alla funzione originaria di meri segnali di anomalia meritevoli di approfondimento». Il testo che ci si propone, sulla base delle modifiche apportate all'emendamento dei senatori Montalbano ed Angius, non tocca l'aspetto strutturale che in quella sede la mozione volle sollevare. Non risolve il problema della eliminazione, per quanto riguarda gli studi di settore, dell'efficacia della inversione dell'onere della prova, ma si limita ad eliminare l'odioso criterio dell'inversione solo per la fase solo per la fase transitoria che precederà la nuova definizione degli studi di settore per la quale è in corso la consultazione con le parti sociali.

che l'emendamento Azzollini ed altri propone, cioè che a regime, definitivamente, per sempre gli studi di settore non producono l'effetto dell'inversione dell'onere della prova

Prego di rendere chiaro ciò che voteremo e di consentire che successivamente all'eventuale approvazione dell'emendamento Angius e Montalbano rimanga per l'Aula

l'attenzione dell'Assemblea sullo scopo delle finalità di questo emendamento, che sono quelle di rendere più chiari, trasparenti e certi i rapporti tra le imprese e lavoratori autonomi e l'amministrazione finanziaria dello Stato attraverso una corretta applicazione degli studi di settore. La questione, come è noto, riguarda milioni di cittadini italiani (commercianti, artigiani e piccoli imprenditori), sui quali - in questo senso concordo con lo spirito dell'intervento del senatore Sacconi - non può, a nostro giudizio, permanentemente pesare il sospetto di evasori fiscali continui. A parte i buoni risultati che sono stati ottenuti, a nostro avviso, dal Governo nel contrasto all'evasione fiscale, oltre che nelle politiche economiche di bilancio - non ho la pretesa su questo di avere il consenso dei colleghi Sacconi e degli altri dell'opposizione però, siamo fermamente convinti che politiche fiscali rigorose esigano un sistema di regole certe ed eque che non possono essere continuamente cambiate, che devono giovarsi nell'applicazione pratica di una amministrazione finanziaria efficiente che garantisca coerenza ed equilibrio nei rapporti con il cittadino ed a questo fine, a nostro giudizio, gli studi di settore muovono in questa direzione. Ora, è ben vero, come veniva ricordato, che anche nei mesi precedenti si è ritornati su questo tema, ne abbiamo discusso anche in Aula di una discussione che abbiamo svolto nel giugno 2007 relativa ad una mozione di maggioranza su questo rilevantissimo tema, abbiamo individuato anche modalità di applicazione degli studi di settore tali da vincolare l'amministrazione finanziaria a dei criteri che non fossero punitivi o coercitivi nei confronti dei lavoratori autonomi. autonomi. Penso, lo dico chiaramente, che probabilmente il Governo avrebbe potuto assumere su questo tema un atteggiamento più aperto ed incisivo e che forse avrebbe potuto accogliere la prima versione dell'emendamento da me presentato con il collega Montalbano, analogo a quello presentato da altri colleghi. Vorrei tuttavia richiamare l'attenzione del collega Sacconi, perché l'emendamento che stiamo discutendo, che mi fa piacere sia stato sostanzialmente condiviso e sottoscritto dal collega Polledri e immagino dai colleghi della Lega, diamo un segnale preciso ai lavoratori autonomi, ma anche al Governo, in merito all'applicazione rigorosa degli studi di settore su un punto fondamentale, che poi è a nostro giudizio essenziale: che l'onere della prova relativa ad un'eventuale disapplicazione, o evasione, se volete, da parte dei lavoratori autonomi, grava sull'amministrazione finanziaria, non sul lavoratore autonomo medesimo.

che, nel momento in cui lei stesso invoca una forma di concertazione per l'applicazione degli studi di settore tra l'amministrazione finanziaria, cioè il Governo, e i rappresentanti delle organizzazioni di lavoro autonomo,

che adesso nella discussione della legge finanziaria dobbiamo approvare una norma strutturale a regime, che dunque valga a prescindere dall'opinione delle organizzazioni autonome. Penso che questo non sia giusto. Invito il

che valgono la presunzione semplice, la non automaticità degli accertamenti e ovviamente» - sottolineo «ovviamente» - «l'onere della prova a carico dell'amministrazione finanziaria». È un passo in avanti

chiesto e ottenuto un'indicazione da parte del Governo molto importante per quanto riguarda le nostre piccole imprese circa, in particolare, la presunzione semplice degli studi di settore e degli indicatori di economicità. Questa riformulazione che è stata proposta dal senatore Angius è un piccolo passo in avanti; sempre un passo è, però sinceramente in questa sede abbiamo assunto altri impegni, come maggioranza e anche come Aula del Senato e come Governo. Governo. Com'è stato ricordato dai miei colleghi, il 26 giugno scorso abbiamo approvato la risoluzione della maggioranza, a prima firma della senatrice Finocchiaro e con la firma di tutti i Capigruppo della maggioranza, in cui si è affermato il principio

gli studi di settore e gli indicatori di normalità economica abbiano natura di presunzione semplice, che non diano luogo ad accertamenti automatici e che l'onere della prova sia da parte dell'amministrazione finanziaria.

che non devono generare accertamenti automatici. Questa è una sicurezza che dobbiamo dare ai nostri piccoli imprenditori, che già si trovano in difficoltà con l'imponente peso fiscale che devono sopportare, e almeno devono avere la certezza che quello che è dichiarato, quello che riescono a generare effettivamente sia il reddito che devono dichiarare e che non sia un reddito fittizio venuto fuori da dati statistici sui quali poi

in prima lettura della finanziaria, riusciamo a dare solo un minimo segnale, che effettivamente avevamo già dato quando abbiamo approvato il "tesoretto", e non riusciamo a dare seguito agli impegni che qui in Aula abbiamo preso rendendo strutturale questa manovra.

Signor Presidente, mi accingo a dichiarare il voto favorevole ad una sola condizione, che vorrei proporre ai presentatori e all'attenzione ovviamente del Governo e del relatore, quella di sostituire le parole: «elementi di prova» con le altre: «le prove», con una definizione quindi più certa e più semplice.

Questa norma, senatore Angius, è invero - diciamocela tutta - ultronea, perché, come ha ricordato la senatrice Thaler Ausserhofer, una disposizione forse anche un po' più coraggiosa era già stata approvata dal Parlamento nell'occasione testé ricordata, perché, se l'onorevole Lettieri ebbe a dire in quest'Aula che gli studi di settore e gli indici di normalità devono avere come conseguenza la presunzione semplice, quindi non l'inversione dell'onere della prova, invece in questo caso ci limitiamo ai soli indicatori di normalità, che concorrono a definire gli studi di settore, ma che sono per definizione, essi certamente, semplicemente lo dice la parola stessa - elementi utili a individuare un'anomalia e nulla di più. Era stato il Governo, erroneamente, ad attribuire ad essi l'efficacia dell'inversione dell'onere della prova, ma avevamo già chiarito, fortunatamente, in quest'Aula che gli indicatori di normalità devono servire solo a quello, cioè solo a selezionare gli accertamenti, nulla di più. Peccato che, invece, nella mozione della stessa maggioranza, nelle dichiarazioni della sottosegretario Lettieri e ovviamente nella tesi dell'opposizione si fosse detto che il complesso sistema degli studi di settore doveva dare luogo al superamento dell'inversione dell'onere della prova: è questo ciò che manca nell'emendamento che stiamo esaminando. Non possiamo che essere d'accordo, a questo punto, nel votare a favore dell'acqua fresca, perché un bicchier d'acqua non si nega a nessuno, ma nella consapevolezza che il problema rimane tutto. Rimane, cioè, il problema dell'intollerabile conseguenza di uno scostamento dallo studio di settore. Anche dopo che gli studi di settore verranno concordati - ci auguriamo - con le organizzazioni di tutela e rappresentanza del lavoro autonomo, rimarrà in piedi l'odiosa conseguenza dell'inversione dell'onere della prova: di questo ci lamentiamo, questo contestiamo. Peccato che poco fa l'Assemblea non abbia voluto approvare l'emendamento del collega Azzollini ed altri, che questo prevedeva. Pertanto, con questi limiti e con la proposta che abbiamo fatto,

e dalla senatrice Thaler Ausserhofer. È evidente che si tratta di una misura transitoria, tuttavia, anche sulla base della mozione che abbiamo discusso e degli impegni assunti dal Governo, vi è in corso

per due ragioni fondamentali. In primo luogo, esso conferma una certa coerenza al rispetto della prassi del contenzioso tributario, che è fondato da sempre sull'onere della prova a carico dell'accertatore, in questo caso a carico dell'Agenzia.

cioè di norma in attesa di una disciplina di riforma organica (più organica) di questo settore, allora percorriamo strade più compromissorie e più attenuate; ogni norma è transitoria e suscettiva di successive integrazioni e modificazioni. Quindi, noi riteniamo, in coerenza con la dottrina del contenzioso tributario e in coerenza con la consuetudine finora applicata in termini di accertamento, che il nostro emendamento, al pari di quello del collega Angius, debba avere grande approvazione; anzi, auspico

vi è opposizione a questa richiesta di modifica per una ragione sintetica: questa disposizione incide sulla fase di accertamento, come è scritto nella norma stessa, nella quale l'ufficio non può che fornire elementi di prova, non prove definitive, le quali vanno acquisite nella fase dell'accertamento definitivo, ovvero del contenzioso, da parte del giudice tributario. Pertanto, non è possibile apportare questa modifica perché implicherebbe la valutazione di problemi molto complessi che rimetto al Governo. Governo. Gli elementi di prova dipendono da fattori di varia natura; la prova vera e propria è un elemento che non sempre è disponibile. Il contenzioso e la discussione sono fatti sulla base degli indicatori, ma, evidentemente, anche sulla base della costruzione di una dialettica con il contribuente. questione in questi termini significa creare un forte indebolimento e aprire un problema serio di gettito. Invito quindi il proponente a mantenere il testo originario, che riceve l'accoglimento del relatore e del Governo.

Presidente, come dicevo, parliamo di una distinzione molta tecnica tra "elementi di prova" "prova". L'attività dell'ufficio, nei confronti della quale questa norma pone delle regole...

l'ufficio acquisisce elementi di prova, valutazioni che riversa nel verbale di accertamento; dopodiché, nella fase definitiva dell'accertamento, ovvero nella fase del contenzioso, viene acquisita la prova definitiva. Questa norma, quindi, incide nella fase preliminare, in cui si attiva l'accertamento tributario. Ecco perché non vi può essere, allo stato (a meno che le mie argomentazioni vengano smentite sotto il profilo tecnico), una valutazione positiva su questo testo. Signor Presidente, mi scusi, ma ma la norma che stiamo per approvare o è acqua fresca, come sosteneva il senatore Sacconi, o non lo è. Secondo me, non è acqua fresca, perché questa norma, rispetto al testo del decreto

luogo, differisce nel tempo, fino alla formulazione dei nuovi studi di settore, l'efficacia della norma. Siccome è una norma importante, non vorrei che per questa frettolosa

il presidente Angius a rivedere la sua posizione. In caso contrario, sulla base delle valutazioni e acquisizioni che avevamo fatto in precedenza, dovrei esprimere un parere contrario. Ma non lo voglio esprimere, il parere contrario. Quindi, chiederei

È del tutto evidente che quando maneggiamo una materia che interessa questi importi dobbiamo muoverci con grandissima attenzione: basta un parola, una virgola per modificare la struttura della questione. Allora, se - come mi auguro e invito a fare - il presidente Angius mantiene il testo precedente, e lo prego vivamente di farlo, di farlo, il Governo lo accoglie, anche se forza molto il ruolo degli indicatori provvisori, mantiene in modo molto forte la concertazione con le categorie che qui è richiamata i nuovi studi di settore sono frutto - e il Governo si è impegnato a farlo anche con un comunicato - della concertazione, quindi usciranno dal confronto con le categorie. Se questo, però, non dovesse essere, sono costretto a chiedere l'accantonamento, non posso non chiedere la relazione tecnica, compresa la bollinatura della Ragioneria dello Stato, e sono purtroppo certo che alla fine sull'emendamento facciamo una frittata, cioè rischiamo di non poterlo approvare perché stiamo parlando di cifre che si moltiplicano con grande immediatezza. Ecco perché in modo molto accorato - lo dico con grande sincerità prego il presidente Angius di mantenere il testo precedente. una richiesta di accantonamento non si nega mai, per carità;

presentato dal senatore Angius, che prevede una copertura, è evidentemente ammissibile anche se il Sottosegretario ha accennato a difficoltà di copertura, mentre l'emendamento di cui è primo firmatario il senatore Polledri, che è stato reso ugualmente ammissibile, non prevede alcuna copertura. Ergo, se ne deve dedurre che la Presidenza

- statuito dalla Presidenza che non c'è onere. Anche il Governo dovrebbe mettersi d'accordo con se stesso, o comunque con la Presidenza del Senato. Se è vero che non c'è onere, non vedo perché non si debba votare al momento. Senatore Castelli, i due emendamenti sono identici, i due presentatori si sono orientati nello stesso modo. Ora, non stiamo discutendo nel merito, c'è la richiesta di accantonamento che non tocca il merito. Il proponente Angius è d'accordo nel metterli un momento da parte, quindi, il risultato della combinazione dei due emendamenti può anche non cambiare. Credo che si potrebbero accantonare tutti e due. Presidente, gli emendamenti sono due, c'è un titolare che è il senatore Angius e c'è un titolare che è il senatore Polledri, che ha delegato a me, in qualità di Capogruppo, l'ingrato compito di prendere una decisione (d'altro canto i Capigruppo servono per questo). I due emendamenti, anche se sono identici nel disposto, non sono identici del tutto perché nella versione del senatore Angius sembrerebbe che l'emendamento

il senatore Angius e togliere il Governo e la maggioranza da questa ambascia. Chiusa la parentesi, dicevo che questo emendamento prevede una copertura e la trova,

tecnico-politica è che il senatore Angius non si è pronunciato, ma ha chiesto solo un momento di riflessione. Questo è il dato di fatto.

a quello esposto dal relatore Legnini. Mutare l'espressione "elementi di prova" in "prove", lo dico ai molti giuristi presenti, non è un elemento garantista per il contribuente, perché è nel contraddittorio che si instaurerà tra l'Agenzia delle entrate e il contribuente che gli elementi di prova

Ho accettato, come è stato proposto dal Governo e dal relatore, la proposta di accantonamento esattamente per quelle motivazioni espresse dalla senatrice Finocchiaro e da ultimo dalla senatrice Rubinato. Qualora, però, si decidesse di procedere al voto

Mi sembra che l'intervento del senatore Angius abbia chiarito la questione: egli è disposto a votare la stesura originaria dell'emendamento

a tutti coloro che operano, anche a livello imprenditoriale, nel settore forestale, ma esclusivamente alle società cooperative, cioè alle imprese collettive che perseguono finalità mutualistiche, equiparandole quindi, ai fini del regime agevolato IRAP, anche alle cooperative della piccola pesca, della mutualità e della marginalità territoriale. Quindi, ritengo opportuno evitare, con l'approvazione di quest'articolo, una lesione di *par condicio* fiscale che mi sembra ovvia e che sarebbe ingiusto non applicare.

**Il Senato non approva.** colleghi, se possibile, vorrei attirare un attimo la vostra attenzione, perché qui si propone la soppressione di un

Di cosa stiamo parlando? Di una misura che prevede che una quota parte delle entrate recuperate dalla cosiddetta evasione fiscale venga distribuita tra il personale del Ministero delle finanze. Questo ha comportato due gravi patologie. La prima è che si introduce una sorta di conflitto d'interessi, perché è evidente che nell'accertamento colui che accerta sa che maggiore sarà l'accertamento, maggiore sarà probabilmente la gratifica che gli verrà data a fine anno. La seconda devo dirla, perché forse è una notizia che è stata tenuta riservata per troppo tempo: la conseguenza la conseguenza pratica di tutto ciò è che nel 2005 il personale del Ministero delle finanze si è distribuito e suddiviso 800 milioni di euro a mo' di gratifica

Credo che abrogare questa norma sarebbe un esempio di etica ed anche di calmieramento degli stipendi di alcuni funzionari statali che raggiungono cifre

anche quello che accadde nel 2005: arrivò in Consiglio dei ministri la denuncia del «Corriere della Sera» (fu Gian Antonio Stella a scrivere e denunciare lo scandalo in questione). Ora, ricordo una discussione molto accalorata in Consiglio dei ministri: l'opposizione di allora scrisse comunicati di fuoco contro il Governo del Paese, che tollerava quello che si definiva uno scandalo; vi furono prese di posizione, colleghi, dei sindacati ministeriali degli altri Ministeri che denunciavano la disparità di trattamento. Questo è un privilegio che dobbiamo cancellare, signor Presidente: approvare questo emendamento significherebbe dare un segnale di moralità alle istituzioni, perché esso restituisce quattrini alla collettività. Spero che il Ministero dell'economia dia un parere favorevole, perché ciò vorrebbe dire mettersi in sintonia con le attese della pubblica opinione. Non togliamo un euro alla politica (e già di per sé questo non è bello), ma almeno togliamo risorse immotivate a chi è pagato già di suo per fare il proprio dovere.

dall'esistenza di infrastrutture aeroportuali così ingenti. Abbiamo pensato di ricavare, senza oneri aggiuntivi per la pubblica amministrazione, un *quantum* limitato per tutti i biglietti di ingresso finalizzato al supporto delle popolazioni per la realizzazione di infrastrutture.

Signor Presidente, esprimo su questo emendamento delle brevissime osservazioni

alla estensione delle sale da gioco sul territorio nazionale ed all'installazione nelle sale Bingo e nei locali collegati delle *slot machine*. Alcuni di noi sono anche presentatori di un disegno di legge sulla patologia da dipendenza. Ci teniamo, quindi, ad evidenziare che questo problema non deve essere sottovalutato da parte dello Stato, sopratutto per le responsabilità che lo Stato ha da questo punto di vista. Quindi, chiediamo al Governo d'individuare una fonte di entrata diversa rispetto a questo e ci impegniamo come Parlamento ad affrontare il problema dal punto di vista legislativo e chiediamo al Governo di collaborare in tal senso, ma soprattutto, di individuare delle risorse da una fonte diversa. Siamo profondamente convinti che lo Stato deve, in ogni caso, assumere responsabilità di assoluta trasparenza. Ci sembrava corretto evidenziare questo di fronte all'emendamento sul quale comunque noi, non essendo la sede idonea, esprimeremo un parere contrario.

mi pare il decreto Bersani-Visco - aveva presentato un ordine del giorno sulla materia al posto di un emendamento. Il senatore Polledri sa che quell'ordine del giorno non è rimasto senza seguito perché poco dopo, anche sulla base della delega che avevo ottenuto, ho scritto ai Monopoli di Stato perché si attenessero alle indicazioni dell'ordine del giorno e del Parlamento. Credo che abbia ragione la senatrice Baio che ringrazio perché questa non è la sede per risolvere il problema. Se il senatore Polledri volesse trasformare questo emendamento in ordine del giorno, l'impegno del Governo ad affrontare il problema c'è, anche se in questo momento non ho disponibile la soluzione immediata. Ringrazio la collega ed il Sottosegretario del garbo. Faccio presente, Sottosegretario, questo sarebbe il quarto ordine il giorno che approviamo sull'argomento. Il primo, a firma di Gianluca Pini, presentato il 2 agosto 2006, che più o meno chiedeva di trovare una soluzione;

Potrei anche dire al sottosegretario Grandi - ma non voglio infierire perché lei sa che potremmo farlo - che ci sono oggi delle storture che attengono alla alla commistione (abbiamo fatto un grande parlare di commistione di interessi, magari del presidente Berlusconi)

attenere anche ad alcune strutture politiche vicine alla maggioranza. Oggi però, lo dico con molta pacatezza, credo non si possa rimandare. Ringrazio dell'invito, ma, in coscienza, non si può rimandare. Non ci sarà mai una sede, signor Sottosegretario, e in politica molte volte bisogna avere anche il coraggio delle azioni. In merito, rivendico con orgoglio

Nella discussione di questa proposta emendativa si è più volte fatto riferimento, a partire dalla senatrice Baio e poi anche dai rappresentanti dal Governo, al fatto che la finanziaria non sarebbe la sede la sede adeguata. Probabilmente, mi sono distratto nella discussione, ma non so se ci siamo accorti che stiamo parlando di una serie di emendamenti che aggiungono norme al comma 74 dell'articolo 5. Sono andato a leggere quello che dice il Servizio studi di questa istituzione, il Senato della Repubblica,

del 20 aprile 2001, articolo 3, lettera c)) l'introduzione, con legge", - come fa questo comma - "di una modifica frammentaria in una fonte non avente forza di legge". Il Servizio studi dice che il comma uscito dalla Commissione alle normative previste dalla circolare del Presidente del Senato. Qui si sostiene che non è la sede, mentre il Senato dice che non è così che si fanno le leggi. Vorrei allora capire due cose: in primo luogo, se dobbiamo andare avanti con la votazione di un comma

vuol dire che i colleghi Baio e i rappresentanti del Governo devono chiedere scusa al senatore Polledri, dicendogli: "Abbiamo sbagliato; poiché pretendevamo di far votare norme che non sono conformi, adesso votiamo anche il suo emendamento". Altrimenti, non credo che si possa uscire da questo bivio.

obbligatoriamente, la seduta di lunedì è ridottissima e la sola giornata di martedì avrà i tempi completi. Se vogliamo procedere all'esame degli articoli e votarli,

Presidente,questo emendamento pone una questione drammatica Lo so che a voi non importa niente della povera gente che si vede espropriata la propria abitazione per un credito inferiore ai 10.000 euro. So benissimo che a voi di queste cose non importa niente, perché si tratta di questo. Forse non l'avete capito perché non avete letto i giornali e non vi siete interessati ai problemi di quanti si vedono espropriare espropriare la propria abitazione per crediti inferiori ai 10.000 euro, soltanto perché i concessionari ormai si comportano peggio degli usurai.

*(FI)*. Signor Presidente, l'emendamento 6.6, sottoscritto anche dal senatore Vegas e dal senatore Ferrara, riguarda la metropolitana di Torino e di Palermo. Nella discussione del decreto‑legge il Governo si era impegnato, a fronte della della soppressione dell'emendamento che avevamo presentato per coprire lo stanziamento delle metropolitane di queste due città, di assolvere a tale impegno durante la finanziaria.

segnalare all'Assemblea la necessità di evitare quella che può apparire alla lettura del testo un'autentica presa in giro. Con l'emendamento 6.10 proponiamo di sopprimere al comma 5 la lettera *c‑bis)* che è stata introdotta.

acquistare elicotteri destinati ad un servizio minimo di trasporto pubblico locale per garantire collegamenti con le isole minori nelle quali esiste un fenomeno di pendolarismo. È giusto, ci sono isole minori (questo tema è riecheggiato spesso nell'Aula), quindi per chi vuole andare in continente con l'elicottero ci deve essere la disponibilità da parte delle istituzioni ad aiutare le persone. Quale è il problema che solleviamo, e per questo proponiamo l'eliminazione di quel comma? Lo dico per una ragione di serietà nei confronti dei cittadini di quelle isole, anche perché

che stanziava 100 milioni di euro (2007, 2008 e 2009) per far sì che i cittadini avessero un servizio di trasporto pubblico

devono essere sottofinanziati, oppure si fa cosa seria se si aggiungono risorse per acquistare gli elicotteri. Con questa misura sottraiamo dunque risorse al trasporto pubblico locale, che abbiamo sostenuto con la legge finanziaria dell'anno scorso, e illudiamo i cittadini delle isole minori che ci siano risorse per acquistare gli elicotteri. Questa è un'autentica presa in giro che credo il Senato non possa far passare.

Roma, Milano e Napoli per lavori relativi a un miglioramento del trasporto pubblico locale. In quel caso, noi avevamo proposto emendamenti tendenti a redistribuire le risorse, che erano pari a 500 milioni di euro, a favore della città di Roma, in modo tale da favorire quelle disponibili per gli enti locali

talché la possibilità di risorse per la capacità di imposizione locale era bastevole, secondo le nostre valutazioni, a recuperare le risorse da

dal Governo in Aula e supportato dalla maggioranza che aveva votato contro il nostro emendamento. Mi riferisco all'individuazione di risorse per quei sistemi che appartengono da un lato a Torino, che ha bisogno di sviluppare enormemente la possibilità di un trasporto pubblico più efficiente, e dall'altro lato a Palermo, altro caso in cui addirittura c'è una progettazione esecutiva, con la possibilità di andare in appalto e di individuare il *general contractor*. C'è una difficoltà ad individuare le risorse necessarie che la misura minima, la progettazione esecutiva, ha individuato come tali.

iscritta nella logica del "si dice, ma non si fa". Ecco il motivo per cui dichiariamo il nostro voto favorevole all'emendamento 6.6 e vorremmo recuperare alla nostra proposta tutti i

enormi, incredibili, che hanno un significato specifico soltanto nella natura altamente politica della gestione della cosa pubblica a Roma e nel Lazio. Ci si deve rendere conto che non si può fare politica con i soldi degli italiani; si dovrebbe capire che queste sono cose importanti, per cui un "sì" può migliorare la nostra capacità di disporre leggi che abbiano un significato vero e non quello politico, e mistificatorio a cui la vostra logica finisce per appartenere. Ma non è la nostra logica: noi voteremo a vostro favore e speriamo ancora che qualcuno di voi si possa

Ma noi dobbiamo dire ai cittadini le cose come stanno. Lo scorso anno avete stanziato con la finanziaria 100 milioni di euro ‑ ho trovato finalmente la norma ‑ per acquistare veicoli ferroviari, nella misura massima del 75 per cento, per l'espletamento dei servizi ferroviari di interesse regionale e locale, per i servizi ferroviari di interesse regionale e locale in concessione, per veicoli destinati a servizi su linee metropolitane, tranviarie o ferroviarie, per autobus a minore impatto ambientale.

un termine caro al Ministero dell'economia). Ebbene, vorrei che si evitasse la presa in giro dei cittadini. Credo che sia una domanda legittima, che ci sia il dovere di rispondere da parte del Governo

sulle quali, se ci si vuole impegnare per investire, si possono prevedere più risorse: non si spendono gli stessi soldi dello scorso anno per acquistare cose che lo scorso anno non erano previste.

L'articolo 6 destina risorse cospicue - circa 500 milioni di euro - per le nostre città, per migliorare il servizio ai cittadini, migliorare i mezzi e le reti di trasporto collettivo; produce anche una forte innovazione con la defiscalizzazione degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale, una novità chiesta da molto tempo e che finalmente trova una soluzione. Voglio anche sottolineare che queste risorse, pur significative, sono riferite soltanto all'anno 2008, quindi non hanno quel carattere strutturale e stabile che la situazione del traffico dei pendolari e del trasporto nelle nostre città richiederebbe.

Naturalmente, conosco bene il carattere solo esortativo di un ordine del giorno, ma ricordo al Governo soprattutto, oltre che alla maggioranza e all'opposizione, che presso la Presidenza del Consiglio è stato istituito un tavolo con le Regioni, le imprese di trasporto e le organizzazioni sindacali, che ha proprio concordato sulla necessità di sviluppare e sostenere il trasporto collettivo anche nell'ambito della riforma dei servizi pubblici locali con risorse strutturali. Una risposta strutturale in questa finanziaria e in questo ramo del Parlamento non è stata ancora identificata e per questa ragione il settore ha indetto per il 14 novembre una giornata di mobilitazione, che naturalmente ci vede attenti e proprio interpreti di questa esigenza. Con la mia dichiarazione di voto a favore dell'articolo 6, un articolo importante, vogliamo però anche sottolineare la necessità di trasformarlo in una misura strutturale

all'ipotesi di credito di imposta già disciplinata dal testo altre ipotesi relativamente agli utili delle imprese produttrici ed altre norme utili che si commentano da sé.

un principio fortemente innovativo, parzialmente già contenuto nel testo della finanziaria presentato dal Governo per quanto riguarda, come è noto, il credito di imposta. Qui si fa qualcosa che, a mio avviso, è ancora più liberale, cioè si parla della detassazione degli utili reinvestiti nell'impresa per scopi che sono dichiaratamente di carattere culturale. In questo senso, ci allineiamo

alla produzione italiana e alla sua circolazione. Sappiamo che la produzione italiana, anche quando attinge livelli di qualità, spesso non riesce a farsi conoscere perché la distribuzione privilegia di gran lunga i prodotti che fanno cassetta o che hanno già un *background* di critica favorevole.

Sostanzialmente ci riferiamo a quelle più tradizionali e non alle multisale che ormai fanno parte dei circuiti di grandi multinazionali.

un uomo di cultura liberale. Vorrei sapere come si fa a pensare di utilizzare uno strumento finanziario per introdurre una discriminazione sulla qualità culturale della produzione. Avrei paura di vivere in un Paese in cui si finanzia o non si finanzia una produzione artistica a seconda che abbia un tema trattato in un modo piuttosto che in un altro. La libertà artistica e creativa deve essere garantita e, da questo punto di vista, la formulazione del testo mi pare ineccepibile.

che pur svolgono attività che a volte sono direttamente e assai più profondamente utili ai cittadini e che devono pagare le tasse. Questa è veramente una piccola mancia che si dà un settore che fa parte dell'egemonia culturale della sinistra e che deve perciò finanziare con questo piccolo provvedimento.

del mio intervento. Il settore da tutti è dichiarato delicato e in difficoltà. Oggi con questo emendamento possiamo offrire qualcosa al settore cinematografico

lo dico ai colleghi ‑ che punta a far risparmiare o a far investire in cultura chi impiega risorse proprie nella produzione e nella distribuzione dei film. Non concorre a formare il reddito imponibile l'utile dichiarato dalle imprese italiane operanti in settori diversi da quello cinematografico e li impiega nella produzione e nella distribuzione. Credo che questo sia un argomento al quale prestare la massima attenzione. Questo è il motivo per cui ci dichiariamo favorevoli all'approvazione dell'emendamento 7.5 (testo

che trovino anche un riscontro nel mercato, sono disposto ad esprimere un voto favorevole, con una sospensione del giudizio, per vederne poi l'applicazione.

a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte dirette gli utili dichiarati dalle imprese di produzione e di distribuzione cinematografica...», poi reinvestiti. tratta di utili reinvestiti, ma come possiamo, in sede di finanziaria, non approfondire per qualche minuto questa questione e consentire al senatore Bordon di riscrivere il testo in modo corretto? È solo una proposta: un accantonamento per migliorarne il contenuto tecnico.

Proprio per questo, si rende ancora più urgente e necessaria una legge che dia ordinamento chiaro a tutto il sistema cinematografico, indicando cioè come selezionare le aziende a cui dare i contributi e istituire forme di mutualità tra il cinema e la

il concetto che ho sinteticamente formulato in sede di espressione del parere: com'è noto a tutti i colleghi, il testo della finanziaria contiene l'introduzione di un credito d'imposta per le imprese non del settore cinematografico,

estendere tale beneficio fiscale alle imprese produttrici cinematografiche e della distribuzione, detassando gli utili.

Credo costituisca un elemento di cognizione comune il fatto che queste imprese ricavano utili in misura molto limitata. Quindi, è un intervento che perfeziona e integra il testo, nella logica di favorire non un'azienda, ma il cinema italiano. Questo è uno degli

In questa finanziaria, il Fondo per lo spettacolo viene ulteriormente aumentato. Si dice che vi è bisogno della ricerca, della competitività, delle infrastrutture; i soldi, però, sono sempre per i nani e le ballerine. evidentemente, dev'essere il primo effetto di Veltroni segretario del Partito democratico: si vogliono dare ulteriori soldi. La Lega, ovviamente, si sottrae a questo giochetto: preferiremmo che tali fondi venissero destinati ad esigenze più serie, perché questo ci fa prefigurare quale sarà il Governo con Veltroni come Primo Ministro: notti bianche, balli, canti, festival; ma ricerca e quant'altro, zero.

Abbiamo invece tagliato su alcune voci che riguardano in particolare la giustizia amministrativa (Consiglio di Stato, assunzioni a dismisura e, in particolare,

del comma 2, della lettera *f)*, e dei commi 4, 7, 10, 13 e 14, mentre salviamo tutta la parte che riguarda la Guardia di finanza, che riteniamo indispensabile per esercitare un'azione di controllo sull'evasione fiscale. PRESIDENTE.

senatore Turigliatto,

la possibilità di rimborso per attività di riunioni relative ovviamente all'attività parlamentare con rimborsi documentati, a pie' di lista, e comunque entro tetti ben precisi. Introduce, inoltre, un'altra condizione completamente diversa per i cosiddetti portaborse, nel senso che è facoltà del parlamentare indicare una persona di fiducia che lo assista nel proprio lavoro. Tale persona

modifica sostanzialmente la questione del vitalizio, abolendo la possibilità di una pensione particolare con riferimento

alcun ente previdenziale, viene costituito o indicato un apposito fondo. E' chiaro che se fosse approvato questo emendamento si darebbe una risposta molto forte rispetto alle attese e ai costi della politica e anche al discredito che i parlamentari hanno per i loro privilegi, che sappiamo essere assai importanti.

ovviamente siamo contrari all'emendamento del senatore Turigliatto, pur comprendendone le ragioni. Inviterei il senatore Turigliatto, Franco, a considerare l'impegno grande che vi è stato a che la battaglia contro i costi impropri della politica, a cui sicuramente si rivolge questo tema, avesse centralità in questa finanziaria. Penso, ad esempio, al tema del limite stipendiale introdotto, sul quale ovviamente vi è una discussione, ma dove il principio di fondo è stato dal senatore Turigliatto citato in un precedente intervento. Nessuno può mai guadagnare più di dieci volte un salario operaio medio. Quel che, però, voglio rilevare è che in questa vicenda, vi è un'iniziativa presa dai due Presidenti di Camera e Senato e dai questori, tesa effettivamente a ridurre fortemente le prerogative dei parlamentari, sia dal punto di vista presidenziale sia dal punto di vista dell'indennità. Infatti, in questa finanziaria troviamo una soluzione affinché l'indennità del parlamentare sia bloccata almeno per cinque anni. In secondo luogo, credo sia sbagliato dare il senso che il tema principale dei costi impropri della politica sia la retribuzione del parlamentare. Ecco perché, come vi è stata giustamente una discussione che continua sul protocollo del *welfare*, è giusto che si modifichino alcuni aspetti pensionistici rispetto ad una serie di prerogative. Ma quel che non consideriamo giusto è che, in un momento nel quale siamo quelli che ancora sentono viva l'onda di partecipazione che per quel che ci riguarda il 20 ottobre scorso ha portato migliaia di donne e uomini a Roma, è su quel terreno che vogliamo garantire al parlamentare la libertà di azione. È noto, peraltro, che le forze che si richiamano al movimento operaio e comunista giustamente finanziano il partito, anche con le loro indennità. Ma non è questo il tema principale. Ecco perché riteniamo che è bastato porre la questione di una serie di oneri impropri, legati a stipendi, società miste e ad altre forme dirette e indirette di organizzazione dello Stato, che si è visto dove stanno i veri privilegi. Questo, quindi, cui invitiamo il senatore Turigliatto a ritirare un emendamento del genere, a meno che lo scopo principale di esso non sia quello di una norma manifesto, e a collaborare con noi nella gestione di una iniziativa in finanziaria che, riducendo gli emolumenti a livello locale, contribuendo ad abbassare il tetto massimo dello stipendio in rapporto al presidente di sezione della Corte di cassazione e, più complessivamente, contribuendo, in maniera come mai non era avvenuta, a ridurre i costi impropri della politica, fa un'operazione. Vorrei concludere con un numero: il Governo, al di là dei propositi con il cosiddetto disegno di legge Santagata, è arrivato al Senato senza una riduzione se non del numero dei consiglieri comunali, che a noi non sembrava un problema di costo della politica, ma una risorsa della democrazia. Con l'iniziativa unitaria della sinistra e di tutta l'Unione in questo momento c'è un taglio al di sopra di 400 milioni di euro. Di questo vogliamo discutere ed è per questo che pacatamente, chiedendo al collega Turigliatto un ritiro, in ogni caso annunciamo, se l'emendamento fosse mantenuto, il voto contrario.

controversie interpretative sulla natura e derogabilità delle norme che fissano il livello delle competenze dei parlamentari.

una situazione economica difficile del Paese, soprattutto per l'ampiezza del debito pubblico e la sua incidenza nella capacità di essere anche nuovi investimenti, dato il livello di spesa per interessi. In sostanza, il Governo ha ragionato così: così: se c'è un responsabile primo del debito pubblico questa è la classe politica e quindi pare opportuno

coincide, non a caso, con il termine di rientro sotto il 100 per cento del PIL del livello del debito pubblico. Sembra quasi che vi sia un un patto fra la classe politica e il Paese, in cui la prima rinuncia ad una parte dei propri benefici per riparare a situazioni che ha creato negli anni passati. Il criterio del blocco parziale e temporaneo delle retribuzioni o delle indicizzazioni, che poi compare in una serie di emendamenti in parte discussi e approvati,

e con effetti peraltro permanenti, si blocca l'indicizzazione di quello di quello che sarebbe un aumento normale dei livelli pensionistici. Ritengo quindi che si tratti di una norma che, al di là della sua incidenza pratica, ha proprio un significato importante legato alla transitorietà della

Signor Presidente, vorrei fare una breve considerazione sull'articolo 8, sul quale esprimeremo voto favorevole. voto favorevole. Approvando questo articolo, entriamo in maniera incisiva nell'ambito dell'autonomia parlamentare, e anche gli emendamenti presentati dai colleghi andavano in profondità. Decidiamo, in sostanza, quanto guadagnano i parlamentari. Allora, la mia considerazione, dando per acquisito il voto favorevole, vuole andare un po' oltre questo punto, perché noi, come Parlamento, organo costituzionale, abbiamo un'autonomia di qualità e quantità esattamente uguale a quella degli altri organi costituzionali, forse anche un po' più forte, perché è un'autonomia assistita anche da uno strumento qual è il Regolamento parlamentare, che tecnicamente pone una riserva nei confronti della legge. Quindi, se noi oggi stiamo decidendo incisivamente per quanto riguarda il Parlamento, e lo facciamo ritenendo di essere pienamente legittimati come legislatori, vorrei che fosse acquisito da quest'Aula e considerato un precedente conclusivo che possiamo farlo per tutti gli organi costituzionali e di rilievo costituzionale. Noi avevamo presentato un emendamento a tal fine, che limitava l'incremento della dotazione al tetto d'inflazione programmato, c'è stata poi una spontanea dichiarazione da parte dei vertici degli organi costituzionali di osservanza di questo tetto nell'esercizio della propria autonomia, si è deciso di ritirare l'emendamento, ma vorrei che, con questa votazione, si comprendesse bene che si rende chiaro che il legislatore può entrare in quella materia. Non ci sono zone franche istituzionali nei confronti del legislatore sovrano. Questo vuole significare che il Parlamento deve, a mio avviso, valutare e monitorare con attenzione l'andamento della spesa da parte degli altri organi costituzionali e di rilievo costituzionale oltre che della propria (lo dico con il massimo rispetto, ma anche con la massima fermezza); che non ci sono più zone d'ombra, zone riservate, zone sottratte, e che dunque se, nella prossima occasione in cui il discorso si porrà, non sarà stato osservato l'impegno solennemente assunto, questo Parlamento dovrà assumere su di sé la responsabilità e l'onere di deliberare in proposito ponendo i limiti che dovesse ritenere opportuni. Questo lo dico perché rimanga agli atti e perché gli altri organi costituzionali siano avvertiti che questa è una posizione che il Parlamento della Repubblica oggi esprime. *(Applausi Signor Presidente, con i colleghi senatori Morselli e Losurdo, a nome della componente La Destra del Gruppo Misto, annuncio il voto favorevole all'articolo, perché credo che comunque un ulteriore segnale vada dato al nostro popolo. Questo articolo, il quale prevede che per cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge non si applicheranno gli automatismi che riguardano le nostre indennità,

che stabilì che le indennità mensili spettanti ai membri del Parlamento nazionale fossero ridotte nel loro ammontare massimo del 10

L'altoparlante ha segnalato agli onorevoli senatori che era in corso la verifica del numero legale. Mi sono precipitato in Aula e non c'era alcuna verifica del numero legale in corso. Com'è possibile

È evidente che dal senatore Turigliatto mi separa uno spazio enorme dal punto di vista ideologico, ma credo che non credo che non ci sia, invece, nessuna distanza nella buona fede, quando una persona entra in politica pensando di fare cose che complessivamente migliorino lo stato e la qualità della vita delle persone in generale. Ci divide la tecnicalità strumentale per arrivare al risultato, ma credo di saper individuare la buona fede delle persone. In questo senso, se stiamo sulle tecnicalità, non posso condividere completamente il contenuto dell'emendamento del senatore Turigliatto, perché messo così è più che demagogico, è fuorviante. Effettivamente, infatti, nell'immaginario collettivo l'unico costo della politica che tutti rimarcano è quello dello stipendio dei parlamentari. In realtà, ce ne sono molti altri. Trovo scandaloso che, su 500 milioni

lo sapessero nelle assemblee di Mirafiori, probabilmente quando andate a parlare magari un filino si incazzerebbero. Non si può avere il doppio del costo alla Camera; costo alla Camera; non si può avere il Quirinale che spende il doppio della regina Elisabetta; non si possono avere amministratori pubblici che lavorano diciotto mesi alle Ferrovie e vengono

effettivamente voi siete la sinistra; addirittura Turigliatto orgogliosamente è della sinistra radicale; il collega Villone che è intervenuto è della sinistra estrema: come fate a dire le cose che dite? Voi dovreste rappresentare gli operai e l'80 per cento degli operai prende 1.100 euro al mese. Non credo che quello che dice il senatore Turigliatto sia così sbagliato nella sostanza, soprattutto detto da voi. Gli emolumenti attuali della politica non sono certo l'unico costo della politica, ma nella vostra logica dovrebbe essere un discorso portato avanti con forza. Sento interventi biascicati, in cui non ho capito neanche cosa avete detto, per giustificare che quello che dice Turigliatto non ha senso: perché non ha senso? Ridurre drasticamente lo stipendio dei parlamentari sarebbe un segnale così negativo per il Paese? O forse non volete che il resto del Paese, il popolo, sappia effettivamente le cose che succedono nei Palazzi? Non sanno, per esempio, che il Veltroni di turno, che va in televisione a fare il salvatore della Patria, è già in pensione perché è entrato in politica con i calzoni corti, non credo per meriti, ma come tanti altri che sono entrati facendo

paga solo il 10 per cento di tasse; qualcuno ce lo dovrebbe spiegare! Oppure voi, che fate i comunisti, i compagni, i difensori della classe operaia, come mai vi siete riempiti di appartamenti, comprati sì a un milione di euro, ma che ne valgono tre, quattro, cinque o sei, facendo perdere ogni volta 4, 5 o 6 milioni all'erario, cioè all'operaio della FIAT! Quindi, dette tutte queste cose,

ho chiesto la parola per esprimere il mio voto contrario e fortemente contrario - a questa proposta del collega Turigliatto e a tutte le altre proposte analoghe. Presidente, da troppo tempo in questo Paese, accanto a un'indecente demagogia su quelli che sarebbero i costi della politica, nulla si scrive sui costi che la cattiva politica fa pagare al Paese, mentre i costi sarebbero quelli degli uomini delle istituzioni. Da troppo tempo, accanto a questa demagogia, c'è una viltà dei parlamentari che si vergognano dell'incarico che hanno,

che con le nostre decisioni e i nostri voti decidiamo per l'indirizzo politico del Paese e per cifre enormi: quelle delle tasse dei nostri concittadini. È su quello che dovremmo applicare il massimo del rigore per evitare di buttare via i quattrini. Inoltre, per questa responsabilità che avverto ogni minuto in cui esprimo un voto in quest'Aula ritengo che noi abbiamo una retribuzione inadeguata, insufficiente. In quale posto al mondo si ha una responsabilità di questo tipo e si hanno retribuzioni inferiori a quelle di *manager* dell'industria privata o pubblica o della media impresa? Un amministratore delegato di una media impresa guadagna molto più di un parlamentare e tutto questo lo considero normale e giusto in un mondo libero. È indecente l'idea per la quale l'egualitarismo delle retribuzioni debba portare chi ha una responsabilità di questo tipo ad avere retribuzioni uguali a quelle di chi non ha tale responsabilità. È indecente pensare che non ci debba essere selezione e attrazione della classe dirigente. Voglio un sistema politico che paghi così bene chi ne fa da creare la gara per entrarvi tra le persone migliori del Paese e non un livellamento per il quale si entra, magari, per amicizia o perché si è sotto un padrone o sotto una cordata politica. E allora tutta questa manfrina ipocrita sui costi della politica sarebbe molto più seria se si applicasse alle migliaia di miliardi che in questa finanziaria si sprecano, a miliardi che sono stati stanziati dal Governo per comprare le *constituency* dei Gruppi e dei Parlamenti, per fare lo *shopping* del consenso politico di quest'Aula. Basta con la demagogia sui costi della politica. facciamo piuttosto un'analisi seria e vera sui costi che la cattiva politica e questo Governo stanno facendo pagare al Paese. *(Applausi Signor Presidente, chiedo scusa, ma affronto questo argomento con un certo imbarazzo, perché pare che sia estremamente volgare parlare di denaro.

Ad esempio, quando nella precedente finanziaria ‑ non quella del 2007, ma quella del 2006 ‑ si immaginò una decurtazione del 10 per cento dell'indennità dei parlamentari io, pur potendo optare per lo stipendio di presidente di sezione di Cassazione (che è esattamente quello a cui è ancorata l'indennità dei parlamentari), ritenni opportuno

Ma al di là di tutto questo, anche con riferimento all'articolo 8, che impedisce qualsiasi forma di adeguamento agli eventuali aumenti retributivi dei magistrati, ricordo qua un intervento serissimo svolto dal senatore Silvestri. Davvero non riuscirei a dire meglio ciò che in quella occasione disse con grande correttezza il senatore Silvestri, ponendo tutta una serie di problemi raccordati e ancorati all'indennità parlamentare

debba ricevere una indennità ragionevole e congrua, che per l'appunto è stata parametrata su quella del presidente di sezione di Cassazione. So perfettamente che voterete l'articolo 8, ma a questo punto vi devo dire la verità non da parlamentare, ma da cittadino, da magistrato: commetterete un grave errore, perché sicuramente verrete incontro alla demagogia e alla propaganda, a quella forma di antipolitica non più strisciante che pare pervadere il nostro Paese, ma non renderete un buon servizio alla politica. Ma davvero voi ritenete, a fronte di una critica così serrata e continua, spesso demagogica e propagandistica, che ha per oggetto, per l'appunto, le retribuzioni dei parlamentari, che vi salverete e vi laverete la coscienza sostenendo che per cinque anni lo stipendio, l'indennità parlamentare, non verrà adeguata allo stipendio di presidente di sezione di Cassazione? Davvero ritenete che questo passo possa in qualche modo calmare questa ondata di antipolitica? O davvero forse non aveva e non ha ragione il senatore Silvestri

alle ragioni democratiche che si correlano all'esercizio delle funzioni di rappresentanza. So bene che, ad esempio, in accoglimento di un emendamento del senatore Barbato, si è aumentato lo stipendio dei magistrati,

non salverete né laverete le vostre coscienze, non farete una operazione politica e, anzi, vi consegnerete nelle mani dell'antipolitica; sicché l'emendamento del senatore Turigliatto che oggi chiede il 50 potrà essere nella prossima finanziaria seguito da altro emendamento che chiederà il 70, l'80, il 90 che l'indennità parlamentare, cioè l'indennità che sostanzialmente riguarda un deputato o un senatore, sia davvero esagerata rispetto, non so, agli emolumenti di un capo di dipartimento dell'amministrazione,

compreso i rimborsi spese o le spese elettorali, cioè quello che poi - scusate la volgarità - materialmente entra nelle tasche dei parlamentari, allora avete un altro sistema per agire: sulle spese elettorali, intervenite sui rimborsi spese, ma sicuramente non potete intervenire sull'indennità parlamentare, che è correlata esattamente a quelle esigenze di cui parlava il senatore Silvestri. Dico questo Dico questo perché oggettivamente corrisponde al mio pensiero e perché davvero in quest'Aula nessuno mi può tacciare di aver fatto un discorso nel mio interesse personale, avendovi già segnalato che a me resta sempre la possibilità di optare per l'indennità di presidente di sezione di Cassazione e conseguentemente di non subire gli stravolgimenti economici e democratici

ma credo non si possa adoperarlo per un'operazione di accusa di demagogia e fare dell'altra demagogia. Ci rispettiamo reciprocamente e ognuno ha le proprie idee:

non sia facile spiegarlo ad un invalido che ha 243 euro di pensione e non sia facile spiegarlo... Ripeto, ognuno ha le sue idee e cerchi di rispettare quelle degli altri. Parliamo di invalidi che vivono con 243 euro al mese. Parliamo dei poveri, di quelli di cui parla il Papa, di cui parlano i documenti della Sinistra, ma a cui diciamo che non ci sono soldi,

chiudere. Guardiamo tutto, sistemiamo il Paese e poi consideriamo le prebende dei parlamentari. Se uno non se la sente di difendere tutto questo di fronte alla condizione del Paese può sbagliare, ma non va preso in giro.

collega ha ritenuto corretto stabilire una forbice di retribuzione all'interno della pubblica amministrazione, da 1 a 10.

senza nulla togliere alla dignità dei colleghi che hanno detto che all'apice della piramide dovrebbero stare i rappresentanti del popolo. Ebbene, fatto cento la retribuzione di un parlamentare, non troviamo corretto che all'interno della pubblica amministrazione un Ministro faccia la figura del pezzente di fronte ai suoi dipendenti e ai suoi collaboratori che hanno retribuzioni di gran lunga superiori a quelle a lui corrisposte. Stabiliamo, pertanto, Stabiliamo, pertanto, che gerarchicamente, anche a livello di retribuzioni differite, pensioni, vitalizi e così via,

altrimenti, cari Ministri, sarà dura operare in mezzo a dipendenti che se ne "fanno un baffo", dal momento che del resto i politici entrano ed escono

senatore Villone

ambigua ed ipocrita, perché prevede, sì, che si torni ad un Governo snello, ma a partire dal prossimo

per l'entrata in vigore di una legge. Signor Presidente, mi consenta di far intendere il senso di questo articolo che direi tipicamente «veltroniano», perché dice e non dice, dà e non dà, offre e toglie. È un articolo che propone uno scenario invocato da tanti,

rilasciato interviste e redatto articoli: bisogna snellire il Governo. Allora, la Commissione bilancio ha una sua originalissima trovata: snellisce il Governo a partire dal prossimo Governo. il mio emendamento si divide in due parti: la prima contiene una norma secca che riguarda il numero dei Sottosegretari

vorrei soltanto un chiarimento, cioè un'interpretazione autentica, su cosa vuol dire «prossimo Governo».

Paravia, credo che il «prossimo Governo» richieda un passaggio alle Camere, che esprimono la fiducia; quindi, nel caso del rimpasto, non richiedendosi la fiducia, non si può parlare di «prossimo Governo».

8*-bis* è molto importante: stabilisce il fatto che, dal prossimo Governo, com'è giusto, si provveda ad una riduzione del numero dei Ministeri e ad una semplificazione della compagine ministeriale.

quel decreto presentato dal Governo Prodi il giorno stesso del suo insediamento, successivamente convertito in legge. Ora, in quella legge,

con quella legge - credo opportunamente - esso è stato trasferito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Credo, quindi, sia da intendere la norma contenuta nel comma 2 dell'articolo 8-*bis*, che l'abrogazione è limitata alle norme incompatibili con le disposizioni di cui al comma 1. Naturalmente, qui non avanzo alcuna proposta di modifica del testo, così come predisposto predisposto dalla Commissione, semplicemente, chiedo al relatore se conviene con questo tipo di interpretazione, in modo tale che sia coerente anche con la discussione svolta in Commissione,

Presidente, mi sembra che quanto sostenuto dal collega Vitali sia fondato, nel senso che, a mio modo di vedere, non occorre un'integrazione di questa norma per stabilire che il CIPE rimanga in capo alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Tale

nel decreto di cui si chiede l'abrogazione sia nell'emendamento sia nel testo della Commissione vengono abrogate non solo la parte relativa ai Ministeri, ma ma anche quelle che dovrebbero restare in vita. Pertanto, utilmente ha consigliato al relatore di considerare se quell'abrogazione, presente anche nel testo della Commissione,

Mi viene persino il sospetto che il presidente Calderoli, firmatario dell'emendamento, avesse letto il mio emendamento prima di scrivere il suo, ma è una mera supposizione.

sia persino migliore di quello poi approvato in Commissione, testo che io avevo scritto soltanto perché qualcuno si era fatto impressionare dalla possibilità che la norma riguardasse il Governo in carica, cosa che in realtà non era. Siccome lo ritengo un testo accettabile mi mi esprimerò con l'astensione. Voterò invece contro gli altri emendamenti che sono, a mio modo di vedere, troppo direttamente intrusivi nell'organizzazione del Governo.

di cui però, stante forse anche il fatto che il buon Grillo non si sente più da qualche tempo, si sono perse le tracce. Si sono perse per strada tutte le buone intenzioni del Governo. È rimasta soltanto una polpetta avvelenata.

Non so se se vi siete resi conto che con il vostro voto, sopratutto votando contro l'emendamento 5.100, avete statuito questo principio: ci possono essere boiardi di Stato che guadagnano un miliardo l'anno su cui non vi è alcun problema. Invece, i parlamentari devono guadagnare poco. Vorrei ricordare che la norma sullo stipendio che riguarda i parlamentari è stata costruita nel 1912 da Giolitti per un motivo molto semplice: se i parlamentari non hanno, così come vuole la Costituzione un emolumento adeguato, su questi scranni siederanno solamente due categorie di persone: i ricchi e i ladri. Non credo sia questo che voi volete. Allora vi pregherei di valutare attentamente i prossimi emendamenti che verranno alla nostra attenzione domani mattina.